dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili* «Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»

Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero al senatore Vincenzo La Russa, scomparso domenica scorsa nella sua Paternò, in Sicilia. Fratello maggiore del vice presidente Ignazio La Russa, a cui va il mio sentito abbraccio per la dolorosa perdita, Vincenzo La Russa è stato uomo di fine cultura e di grandi passioni: per il diritto, per la storia, per la politica. Avvocato, insigne giurista, scrittore e saggista, aveva ereditato dal padre Antonino, parlamentare del Movimento Sociale Italiano, un forte senso dello Stato e dell'impegno civico. Dopo essere stato consigliere comunale e provinciale a Milano, la città in cui si era trasferito giovanissimo insieme alla famiglia e dove ha trascorso gran parte della sua vita, Vincenzo la Russa era entrato per la prima volta in Parlamento nel 1979 come senatore della Democrazia Cristiana, partito in cui, per carattere, pensiero, ideali e formazione culturale, si è sempre identificato, militandovi sin dall'inizio della sua esperienza politica e diventandone uno dei suoi più illustri esponenti. In seguito allo scioglimento della Democrazia Cristiana, per la quale era stato anche deputato dal 1983 al 1987, aveva aderito al Centro Cristiano Democratico ed era stato eletto nuovamente al Senato nella XII legislatura, nel collegio di Caltagirone-Paternò. In quella legislatura, come neo eletta senatrice di Forza Italia ho personalmente condiviso con lui tanti momenti tra i banchi di quest'Aula. Ne ho sempre ammirato la grande professionalità, lo scrupolo nell'approfondimento degli atti parlamentari, l'inattaccabile coerenza delle idee, l'instancabile disponibilità al dialogo e al confronto, il rigore morale e il fermo rispetto delle istituzioni: doti che contraddistinsero anche il suo impegno internazionale come rappresentante del Senato in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di cui fu anche autorevole Vice Presidente. Con Vincenzo La Russa salutiamo un caro collega, un amico, un autentico esempio di passione civica e politica, vissuta ogni giorno con dedizione, generosità, concretezza e onestà intellettuale. Alla famiglia del senatore Vincenzo La Russa, al vice presidente Ignazio, al fratello Romano, alla sorella Emilia ai loro cari rinnovo la mia personale vicinanza e il cordoglio di tutto il Senato. In memoria del senatore Vincenzo La Russa invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

i rappresentanti dei Gruppi di tutte le aree politiche che hanno voluto farmi sentire la loro vicinanza. Un particolare ringraziamento va al Presidente della Repubblica, che era amico di Vincenzo, che ha voluto onorarmi con una sua personale telefonata, nonché agli esponenti e ai capi dei partiti di centrodestra e non solo. Non tocca a me ricordarlo: l'ha fatto lei mirabilmente. Dico solo, perché a questo avrebbe tenuto, che forse Vincenzo è stato l'unico parlamentare che veniva eletto senza voti familiari: per questo in famiglia lo chiamavamo la pecora bianca e ne era orgoglioso. Era anche un segnale del fatto il nostro fraterno rapporto - chi ci conosce, come Maurizio Gasparri che l'ha conosciuto benissimo, sa quanto eravamo legati - non veniva minimamente scalfito da posizioni politiche diverse. Di questo sia io che Vincenzo eravamo grati

questo non ci impediva di essere non solo fratelli, ma - se si può - davvero molto di più. Grazie a tutti voi.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi mercoledì 24 novembre, ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori della settimana corrente. Il calendario prevede, con sedute fino a venerdì 3 dicembre, se necessario, la discussione del decreto-legge recante misure in materia fiscale e tutela del lavoro. Nella seduta di domani saranno discusse le relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulle elezioni contestate nelle Regioni Campania, Puglia e nella Circoscrizione estero-Ripartizione America meridionale, nonché la relazione sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto. La settimana dal 6 al 10 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni, in particolare della 5a Commissione permanente, sul disegno di legge di bilancio. Per quanto riguarda la settimana successiva, è stato al momento stabilito che l'Assemblea si riunirà mercoledì 15 dicembre, alle ore 16, per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021.

non soltanto per annunciare che i senatori del Partito Democratico voteranno per la conferma del calendario approvato dalla Conferenza ma anche per sottolineare il peso politico di decisioni che non sono solo procedurali, ma che hanno anche una forte valenza istituzionale.

Ma noto che, come sempre, tutte hanno fondamenta politiche e hanno conseguenze politiche. Il calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo ha previsto per domani la definizione di alcune

Questo ricorso all'Assemblea avviene sulla base del principio dell'autodichia, che fa del Senato il giudice dei titoli di legittimazione dei suoi componenti. il ritardo con cui l'Aula affronta questo delicatissimo nodo è veramente impressionante. Per alcuni casi istruiti dalla Giunta l'Assemblea ha ricevuto le relative deliberazioni da più di mesi, senza contare che siamo ormai nella fase finale della legislatura e alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica non definita situazione dei casi pendenti deve essere anche attribuita la mancata ratifica dell'elezione di due terzi Sinora la ratifica dell'elezione di due terzi dei senatori non è stata ancora effettuata. Ora, non entro nel merito dei singoli casi - ne discuteremo domani - ma dico solo che un ulteriore rinvio aggraverebbe di molto la nostra già molto rilevante inadempienza. Io credo, Presidente, che il Senato debba riflettere sul modo con cui noi stiamo esercitando i poteri che l'autodichia gli attribuisce. Ricordo che la perdita dell'immunità parlamentare è stata la conseguenza dell'uso distorto che ne è stato fatto; che la perdita del finanziamento pubblico dei partiti è figlia della misura eccessiva che aveva raggiunto la cancellazione dei vitalizi è dovuta ai gravi abusi che ne sono stati fatti, persino attribuendo una pensione a vita a chi era stato parlamentare solo per un paio di giorni. Io credo che noi dobbiamo stare molto attenti. L'autodichia è un istituto fondamentale della democrazia, posto a tutela dell'indipendenza del Parlamento. Ma, se continuiamo a rinviare le nostre decisioni, dimostreremo di non saperla usare e anche l'autodichia ci verrà levata.

compie delle visite presso i Parlamenti, facendo delle verifiche sulle regole esistenti nei Paesi. L'incontro di questa mattina verteva sulla legge elettorale. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Zanda che questa cosa non sa.

dicendo che la nostra Costituzione all'articolo 66 assegna al Parlamento, in ultima istanza, la decisione sulle contestazioni. Ciò è talmente vero che in un altro caso controverso di questa legislatura un collega

ritiene. Molte delle votazioni avvengono anche con voto segreto. La non decisione impedisce che l'autodichia, che è uno degli ultimi ruoli residui che il Parlamento ha riservato a se stesso, si eserciti. E se un potere, un ruolo, una responsabilità non si esercita, è giusto che la si perda.

andare avanti per poter consentire a tutti i Gruppi di poter partecipare nella loro interezza al tema che riguarda quanto detto dai senatori Gasparri e Zanda.

comunque proseguano i lavori sul decreto fiscale e che quindi le relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

13 articoli da votare con il collegato degli emendamenti e, quindi, abbiamo bisogno di tempo. Riprendiamo a votare alle ore 17,15, in linea con i lavori dell'Aula. Senatore D'Alfonso, pensate di terminare i lavori questa sera? D'ALFONSO *(PD)*. Noi contiamo di terminare, se arriva a frutto tutta l'attività di confronto politico, a sera avanzata, considerando anche la possibilità delle prime ore della notte.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

18 delle 43 soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, pari al 42 per cento del totale, sono state affidate temporaneamente, da lunedì 15 novembre, a funzionari che per poterle dirigere non hanno superato un concorso pubblico, ma hanno risposto ad un interpello e presentato il *curriculum* al direttore generale competente. Del Ministero della cultura (Mic) se ne sono candidati 256 e 231 erano di altre amministrazioni, ma i 18 sono stati selezionati tutti tra gli interni, scelta comprensibile per i delicati uffici di tutela territoriale, escludendo però gli otto dirigenti dello stesso Mic che si erano a loro volta proposti; uno degli otto aveva assunto da un paio di mesi la dirigenza *ad interim* della soprintendenza per la quale ha concorso, ma non è stato scelto e anzi ha saputo di dover rescindere il contratto e liberare l'ufficio il venerdì precedente a quel fatidico lunedì. Quanto ai 18 fortunati, ce ne sono alcuni (pochi, se non pochissimi) entrati da tempo nei ranghi del Ministero e con un *curriculum* di peso che fa sfigurare quelli degli altri. Nella maggior parte dei casi, infatti, sembra che siano stati scelti oculatamente i funzionari meno titolati, quelli con meno esperienza amministrativa e di tutela sul campo, più giovani anagraficamente o per anzianità di servizio della generazione cresciuta nelle soprintendenze specialistiche anteriore alla riforma Franceschini. Oltre ad assicurarsi l'agognato ricambio generazionale della dirigenza, parrebbe che l'eterno Ministro e tutti i ranghi della sua corte non abbiano mancato di orientare alcune scelte del direttore generale Si vocifera, infatti (e ai dipendenti del Mic non è concesso altro, se non al prezzo di gravi sanzioni disciplinari), che nella eletta schiera degli amici di Franceschino, come è stato ironicamente riportato da «Striscia la notizia», siano presenti più di una pupilla del Ministro, dei vertici amministrativi del Collegio romano e dei dirigenti non generali nelle grazie dei primi per risaputi rapporti amicali. Ancora si sussurra sia stato favorito il coniuge di un dirigente di un istituto di credito tra i maggiori del Paese, specialmente vicino al Mic; più di un funzionario, infine, fra i premiati di questa tornata era già noto alle cronache per vicende personali o professionali non edificanti. L'onorevole Franceschini ha respinto con sdegno quelle che nella risposta scritta ad un'interrogazione di chi parla ha definito insinuazioni destituite di ogni fondamento, che sorprende e spiace possano trovare ospitalità negli atti parlamentari; tuttavia la parte sana del Paese e del Ministero che fu dei beni culturali, ben più sdegnati, sorpresi e dispiaciuti di lui, respingono la sistematica disapplicazione dell'articolo 97 della Costituzione fatta dal Mic e la cristallizzazione mediante prassi di comportamenti corruttivi. Si dimetta, ministro Franceschini, in un sussulto di dignità che, se mai fosse, sarebbe l'unico della sua carriera.

Presidente, l'intervento che mi accingo a fare è molto breve, ma tengo particolarmente a questo ricordo e credo che nei prossimi giorni anche l'Assemblea, con la sua guida, non potrà che ricordare che esattamente 150 anni fa si insediava a Palazzo Madama il Senato della Repubblica. Nella lapide alle sue spalle «L'Italia è restituita a se stessa e a Roma, qui dove noi riconosciamo la Patria dei nostri pensieri, ogni cosa ci parla di grandezza, ma nel tempo stesso ogni cosa ci ricorda i nostri doveri». Era Vittorio Emanuele II ed era il 27 novembre del 1871, esattamente 150 anni fa. Senatore Candiani, mi fa molto piacere che lei abbia ricordato questa data, perché ricorderà anche che nel 2018, dove si è svolta la prima seduta, cioè nel cortile interno, io ho scoperto la targa originaria, che era stata modificata e quindi censurata dal partito fascista;

oggi ricorre un avvenimento importante e mi dispiace non essere nella mia Firenze, nella mia Regione per celebrare la Festa della Toscana. Il 30 novembre di 235 anni fa,

a volere una riforma del codice penale. Questa riforma non era sicuramente perfetta; anzi, conteneva imperfezioni notevoli di diritti, sulle quali anche lo stesso Granduca poi ritornò.

diceva che la vita umana ha un prezzo ineguagliabile e che non deve essere toccata, abolendo la pena di morte. È un onore per me, ovviamente, venire da quella terra, che ha tracciato in qualche modo la storia, purtroppo non in tutto il mondo, ma sicuramente in Europa. È lì la nostra storia. Ci sono i nostri valori, ci sono anche i nostri obiettivi. È per questo che oggi, anche se sono in Senato, avevo piacere di ricordare la festa della Toscana, istituita nel 2000, che ricorda e celebra quell'evento, così importante in tema di diritto e di rispetto della vita umana, che ogni anno diventa anche per noi un impegno: un impegno importante, un pungolo, qualcosa che ci deve stimolare a far sì che in tutto il mondo davvero si arrivi prima possibile ad ottenere quella famosa moratoria, di cui l'Italia ovviamente si è sempre fatta portabandiera, affinché la pena di morte sia abolita. Non vi è niente di più importante, infatti, della vita umana, che non può e non deve essere tolta a nessuno. Sono orgogliosa di dirlo in quest'Aula oggi, in occasione di questo anniversario. *(Applausi)*.

anche alla Presidenza del Senato, che so essere estremamente attenta alle prerogative di ciascun parlamentare e verte su due argomenti. una dirigente della Polizia di Stato, che nel 2017 è stata coinvolta in un increscioso incidente, un tentativo di furto.

Inspiegabilmente, il Ministero dell'interno si sta opponendo, nonostante le decisioni del TAR e nonostante le decisioni della propria amministrazione. Questo è estremamente grave. Abbiamo depositato una interrogazione nel luglio scorso: nessuno si è degnato di rispondere. Analoga considerazione vale per una mozione presentata sulla vicenda dei rapporti tra l'Italia, gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita,

In funzione di questo, è stata depositata una mozione, per sanare una vicenda che sta rendendo il nostro Paese ridicolo, in particolare agli occhi

non rientra all'interno delle prerogative del Parlamento e non rientra all'interno delle prerogative di un parlamentare, in particolare su argomenti così importanti.

si rendano interpreti di questa lamentazione grave, che ho ritenuto necessario affrontare oggi in Senato.

Signor Presidente, sabato 20 novembre si è svolta a Rimini, nel riqualificato Giardino della memoria, un'importante cerimonia commemorativa per le 24 vittime della Banda È stato un ricordo molto sentito e partecipato, che vorrei condividere con tutti voi oggi. Ricordo bene il 30 gennaio del 1988, data in cui, di fronte al supermercato Coop, nel quartiere Celle, venne ucciso

ma la paura e lo sgomento di quell'episodio, che sconvolse la comunità, sono ben vivi ancora dentro di me. Fu un'azione terribile, che costò la vita ad una persona, causò molti feriti, tra cui una bambina di nove anni.

è stato restituito alla nostra città, al termine di un restauro, un luogo della memoria in cui sono presenti 24 targhe commemorative e 24 mandorli per ciascuna delle vittime innocenti cadute per la ferocia della banda dei fratelli Savi che, dal 19 giugno del 1987 al 21 novembre del 1994, causò vittime innocenti (24 morti, (24 morti, 102 feriti), compiendo 103 atti criminali per oltre sette anni e mezzo di terrore e sangue che colpirono la Romagna, Bologna e Ancona. Credo che oggi sia importante condividere questa commemorazione e ricordare quel periodo buio e drammatico del nostro Paese. È in atto un processo di digitalizzazione dei documenti per non disperdere e fare luce sui troppi angoli ancora oscuri di questa vicenda, una digitalizzazione che richiede un impegno, ma anche la salvaguardia di documenti che possono dare ancora importanti rivelazioni. Concludo, signor Presidente, citando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha detto: «La memoria è radice della comunità. Fare memoria è condizione affinché la libertà conquistata continui ad essere trasmessa e vissuta come un bene indivisibile».

e della richiesta del Gruppo Fratelli d'Italia di tenere una riunione nella mattinata di domani, ha stabilito che la seduta di domani abbia inizio alle ore 12,30 per la discussione generale sul citato decreto-legge. Conseguentemente, le relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari già previste dal calendario corrente saranno discusse nella giornata di giovedì. **Atti